*(PD)*. Signora Presidente, discutiamo oggi questa mozione finalizzata a scongiurare la crisi e a definire un possibile rilancio dell'aeroporto di Milano Malpensa, presentata da me e da altri 100 senatori

Cionondimeno, la mozione, di cui presentiamo oggi un testo 2, mantiene ancora una grande attualità. In questi quasi due anni molto poco è stato fatto dalle autorità locali e da quelle nazionali per scongiurare il declino dell'aeroporto. Nonostante un profluvio di parole e di promesse da parte dei partiti di Governo, Malpensa è stata sostanzialmente abbandonata al suo destino ed ha dovuto pensare quasi da sola a definire una ipotesi di rilancio e ad affrontare l'onda lunga della crisi economica planetaria che ha investito, soprattutto nello scorso 2009, anche il traffico aereo nazionale ed internazionale. Malpensa, i milanesi e i lombardi aspettano ancora la visita del Governo Berlusconi, invano sollecitata, peraltro a più riprese, anche da Umberto Bossi, che all'esplodere della crisi Alitalia disse, nel suo linguaggio molto colorito: «Eh Berlusconi *l'è un pù incasà*...»; mi consenta di non tradurre, Presidente. «Però, il problema di Malpensa resta», diceva Bossi. «Perché va bene andare a Napoli, ma bisogna anche andare a Malpensa». Noi stiamo ancora aspettando e attendendo la riunione di Governo allo scalo varesino. Per queste ragioni, la discussione di oggi, sollecitata dalla mozione del PD, può essere ancora utile, perché può essere una sveglia al Governo e una sollecitazione a mantenere gli impegni più volte annunciati. Nella nostra mozione non chiediamo altro: mantenete gli impegni che avete preso con i lombardi, per il rilancio del loro principale aeroporto. Riepiloghiamo per brevi note la questione. La crisi di Malpensa è conseguente alla scelta di Alitalia di abbandonare lo scalo come proprio *hub*. La successiva vicenda del salvataggio della compagnia di bandiera è nota e non merita di ritornarvi sopra, se non per un punto: la bocciatura della vendita di Alitalia ad Air France fu motivata anche dall'obiettivo di difendere il ruolo degli aeroporti milanesi. In realtà, le cose sono andate ben diversamente. Abbiamo speso quasi 4 miliardi Il *de-hubbing* ha portato alla cancellazione del 90 per cento dei voli di Alitalia e ad un fortissimo ridimensionamento del traffico merci.

il decremento rispetto al 2007, ultimo anno normale per lo scalo, è ancora più grave. Se nel 2007 erano transitati da Malpensa quasi 24 milioni di passeggeri, nel 2009 il flusso si è fermato a 17,5 milioni 26,5 per cento). Particolarmente pesante è la riduzione dei passeggeri internazionali (meno 6,3 milioni), mentre più contenuto è il calo dei passeggeri nazionali, calati di 51.000 unità. Il cargo perde nel medesimo intervallo di tempo 2007-2009 il 29,3 per cento, passando da 486.000 a 344.000 tonnellate annue.

avrebbe potuto essere ancora più grave se la SEA non avesse operato per recuperare viaggiatori e merci aprendo lo scalo varesino ad altri vettori. L'arrivo di Lufthansa Italia, nel febbraio 2009, è forse la novità più significativa di questi due anni. Smentendo di fatto le dichiarazioni dei dirigenti della nuova Alitalia-CAI, che non hanno reputato profittevole investire su Milano, Lufthansa ha creato una compagnia di diritto italiano, ha collocato a Malpensa una flotta di nove aeromobili, supportata da un *hangar* per servizi di manutenzione, e ha incrementato l'offerta da Milano di rotte nazionali e internazionali, con l'idea di operare anche per le rotte intercontinentali non appena il mercato lo permetterà. Lufthansa è così passata dal 4 al 13 per cento nelle quote di mercato dello scalo. Altra novità significativa è la crescita della compagnia *low cost* EasyJet. Nel 2009 i passeggeri serviti dal vettore inglese su Malpensa sono stati pari a 4,6 milioni, in crescita del 34,7 per cento rispetto al 2008, rendendo lo scalo la prima base europea di EasyJet per passeggeri trasportati.

Nel settore merci l'aeroporto ha acquisito la nuova compagnia Cargolux Italia, che ha consentito alle imprese lombarde di intensificare le connessioni con Hong Kong, New York e il Canada.

Inoltre, la strategia impostata potrà dare risultati solo a condizione che le politiche di settore siano in grado di rimuovere le criticità che tuttora influiscono negativamente sul buon funzionamento dello scalo. Deve essere cioè chiaro, ancora oggi, che il cuore pulsante della nostra economia nazionale, la Lombardia, che da sola vale il 18 per cento del PIL italiano, non è in grado di competere ad armi pari con le altre regioni più sviluppate del mondo a causa della perifericità del suo principale aeroporto. Secondo un recente sondaggio della camera di commercio di Monza e Brianza, il 65 per cento delle imprese lombarde ritiene fondamentale lo scalo di Malpensa per il proprio *business*. Ancora oggi è bene ricordare che i manager del Nord sono costretti ad andare a Parigi o a Francoforte per raggiungere i mercati mondiali e magari anche Le poche connessioni sono operate prevalentemente da compagnie straniere, mentre Alitalia ha spostato su Fiumicino tutti i voli intercontinentali, riducendo perfino la frequenza sulla richiestissima rotta per New York. La stessa città di Milano ha visto in questi anni, complice anche la crisi, molte multinazionali chiudere le proprie sedi, perché la città è ormai ritenuta periferica e poco collegata alle altre grandi capitali economiche del pianeta. L'Expo 2015, infine, ha fondato una delle sue carte vincenti proprio sui collegamenti diretti con Milano attraverso Malpensa. Oggi la revisione in diminuzione delle attese dei visitatori ha nella difficoltà dei collegamenti aerei una delle principali ragioni. È, quindi, a rischio anche il successo di Expo 2015. Dobbiamo, dunque, ribadire con forza che la battaglia per il rilancio di Malpensa è cruciale per la ripresa della competitività del sistema produttivo lombardo. Per queste ragioni, dobbiamo fare ogni sforzo per risolvere i problemi tuttora aperti, che gravano come macigni su Malpensa. Innanzitutto, dobbiamo riaffermare che la missione di Malpensa è quella di diventare un grande aeroporto internazionale e intercontinentale. La crescita del *low* *cost*, pur essendo una buona notizia, rischia però di determinare una torsione degli obiettivi per cui sono stati fatti tanti investimenti. Malpensa, nato per competere con i più grandi scali del mondo, oggi rischia invece di competere con Bergamo per il *low cost*. Persa la partita per diventare *hub* Alitalia, in attesa di capire se si potrà riaprire il discorso con Lufthansa per divenire un *hub* secondario dedicato all'Europa meridionale, è necessario mettere a sistema la pluralità degli scali lombardi: Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari devono essere coordinati secondo il principio della specializzazione e con l'obiettivo di creare sinergie industriali. In questo quadro Malpensa deve essere l'aeroporto *point to* *point* per il traffico internazionale e intercontinentale, con particolare attenzione alla clientela *business*. Questa è la prima richiesta della nostra mozione: definire al più presto un piano nazionale della rete aeroportuale. Tale richiesta sta in cima agli obiettivi del documento approvato dalla competente Commissione della Camera. La seconda questione da affrontare con urgenza è quella dell'accessibilità dell'aeroporto. Più in generale, l'inadeguatezza dei collegamenti degli scali italiani con la rete stradale e ferroviaria costituisce una vera e propria emergenza. È dunque necessario concentrare le poche risorse disponibili sui grandi scali che hanno l'onere di connettere l'Italia col mondo. Tra questi vi è Malpensa.

Queste opere risolverebbero l'annoso problema dell'accessibilità di Malpensa, creando un collegamento diretto con l'Alta Velocità ferroviaria e con la stazione di Milano centrale, sviluppando forme di intermodalità nel trasporto delle persone e delle merci delle imprese lombarde e venete, e rendendo finalmente funzionale il nesso tra i due terminal. Onorevoli colleghi, mi avvio a concludere chiedendovi attenzione per questa mozione che non esprime solo un'opinione del nostro partito, ma, ne sono certo, coglie in pieno le istanze di un territorio, quello della Lombardia e dell'intero Nord, che vuole continuare a svolgere il ruolo di locomotiva dell'economia nazionale - e le notizie di questi giorni credo ne ne sottolineino l'importanza - e può tornare a svolgerlo con successo solo se si superano le criticità che oggi ne ostacolano la competizione internazionale. Malpensa può essere un grande fattore di crescita economica del Paese. Per queste ragioni, vi chiedo il voto per la mozione posta alla vostra attenzione e chiedo al Governo di passare dalle parole ai fatti mantenendo gli impegni assunti con i cittadini e le imprese lombarde.

queste rappresentano circa 770 milioni di euro in indotto propriamente turistico, ai quali si aggiungono altri 350.000 euro derivati dal traffico aereo per motivi di lavoro. La penalizzazione per il sistema lombardo e del Nord in generale rischia di essere rilevante soprattutto per le imprese rivolte al mercato internazionale, in particolare in questo contesto di crisi, con risvolti molto preoccupanti in termini occupazionali. Malpensa, come ha più volte sottolineato il nostro segretario federale, il ministro Umberto Bossi, è il cuore del territorio padano, il crocevia che collega il Mare del Nord con la Liguria, con Genova. Tre corridoi plurimodali interessano direttamente il nostro Paese ed in particolare, come ricordano giustamente anche i senatori del PdL nella loro mozione, su Malpensa passano i corridoi Rotterdam-Sempione-Novara-Genova (Corridoio dei due mari), Lisbona-Torino-Milano-Trieste-Kiev (Corridoio 5) e Berlino-Monaco-Verona-Palermo (Corridoio 1), collocando quindi Malpensa come nodo, cerniera dei corridoi. corridoi. Dobbiamo operare una scelta fondamentale per il rilancio della nostra economia: dobbiamo imparare a fare i nostri interessi, quelli del nostro territorio, il territorio del Nord, e di conseguenza dell'intero Paese, tenendo ben presente che un attacco a Malpensa diventerebbe un attacco al Nord, alla Lombardia, al Veneto, al Piemonte, che sono la vera e propria spina dorsale dell'intero sistema economico del nostro Paese. Ma andiamo per gradi. Perché investire ancora su Malpensa? Prima di tutto, e noi della Lega Nord lo diciamo da sempre, perché è al centro di un'area che costituisce il motore economico dell'intero Paese, con 1.361.000 imprese. Ricordo che l'aeroporto di Malpensa in dieci anni ha rappresentato in Lombardia una risorsa strategica anche per l'occupazione: 100.000 tra occupati diretti, indiretti e indotto, con il 68 per cento dei biglietti internazionali venduti nel nostro Paese. Potenziare i voli intercontinentali lancerebbe l'economia del Nord di oltre 2,5 punti per Declassare quindi questo *hub* comporterà un taglio di 8 milioni di passeggeri l'anno e la perdita di 1.000 milioni di euro. Sono cifre molto importanti.

Il cosiddetto *de-hubbing* subitaneo posto in essere da Alitalia su Malpensa ha visibilmente provocato una perdita per lo scalo di Malpensa di 4 milioni di passeggeri calcolati su base annua, non recuperati da un contestuale aumento di traffico su Fiumicino, con una perdita per il sistema Paese stimabile prudenzialmente in 4 miliardi di euro. Con l'approvazione del piano di *de-hubbing* Alitalia è passata da 1.238 voli settimanali a soli 352. Per quanto riguarda poi i voli intercontinentali, anche in questo caso non ci sono stati incrementi o variazioni dell'offerta di volo. Un anno fa, poi, nell'aprile 2009, con l'inizio della stagione estiva, quella che dovrebbe quindi far registrare il tutto esaurito o quasi, i voli su Malpensa si sono ridotti ulteriormente passando da 201 a 185, per arrivare a settembre 2009 a soli 159, il che significa che in una sola settimana è partito un solo veicolo all'ora. Ma andiamo a toccare il portafogli: come è variata l'offerta complessiva dello scalo di Malpensa? Riferendoci al periodo di tempo compreso tra il 2007 ed il 2008, vediamo che per le tratte domestiche

8.129 tonnellate di merce che non sono state trasportate sui nostri cieli. E credo che solo questi dati debbano servire quantomeno a lanciare una riflessione: siamo il primo Paese per arte e turismo, abbiamo un indice di *incoming* nettamente al di sopra della media, persone che giungono nel nostro Paese dagli Stati immediatamente confinanti e non solo. E noi vogliamo ridurre, dimezzare, quasi annullare una fonte certa di introito e di rilancio della nostra economia? Qualcuno potrebbe forse dire che lo scalo di Malpensa rappresenta un inutile dispiego di forze e di denaro. Questo potrebbe essere vero se i dati, a due anni dall'insediamento di Lufthansa Italia, non dimostrassero il contrario. Solo a novembre 2008 Lufthansa Italia lancia otto nuove destinazioni intercontinentali proprio sullo scalo di Malpensa, oltre a posizionare *in loco* altri sei aeromobili. A febbraio 2009 poi vengono persino inaugurati due nuovi voli per New York e per Chicago, ed il mese dopo ecco collegate Roma, Napoli e Bari. L'andamento del gruppo Lufthansa Italia 2009 rispetto al 2008 registra un evidente raddoppio degli introiti, e quindi dell'utilizzo delle attrezzature, dello scalo, delle tratte proposte. Lo stesso vale per le altre compagnie, le cosiddette *low cost*, come la EasyJet che proprio su Malpensa ha creato una grossa fetta di mercato e che vede, lo scorso febbraio, la compagnia in maglia arancione sfoggiare 17 aerei di base, nove nuove destinazioni già in vendita ed altre cinque che sono tuttora allo studio degli operatori turistici. Infine, ma potrei citare molto altro, vorrei anche ricordare che da gennaio 2008 a marzo 2009 diverse compagnie aeree di Stati stranieri hanno piazzato sul nostro territorio, nel nostro aeroporto padano uno o più aeromobili di bandiera. Significa che il mercato esiste e noi dobbiamo essere altrettanto bravi da cogliere al volo, e scusate il gioco di parole, le incredibili potenzialità che questo rappresenta. Lo scalo di Malpensa è l'unico grande aeroporto a crescere in tutta Europa: da aprile a dicembre è stato infatti l'unico a registrare un aumento del

Soltanto l'aumento del traffico merci sull'aeroporto di Malpensa nel primo trimestre è stato del 39 per cento, l'unico, o forse uno dei pochi, dove la SEA che lo gestisce ha investito il proprio capitale per apporre alcune sostanziali migliorie. Insieme ad una ridefinizione dei percorsi interni ed una ridefinizione dell'offerta commerciale, la SEA ha anche affiancato un vero e proprio *restyling* non solo dell'aeroporto di Milano Malpensa, ma anche di Milano Linate, del Terminal 2 oltre alla realizzazione di due nuovi parcheggi. Altro punto fondamentale, però, è quello legato alle infrastrutture collegate all'aeroporto di Malpensa. Le opere cosiddette connesse, previste dal *dossier* Expo 2015, sono fondamentali, infatti, per il collegamento tra Malpensa e il resto del territorio, atteso che, in tutti questi anni, lo Stato fino ad ora non aveva mai provveduto ad erogare i necessari finanziamenti atti a inserire l'aeroporto di Malpensa in un contesto infrastrutturale all'altezza del suo ruolo di aeroporto intercontinentale. Le opere connesse avviate dal Governo sono sia sul fronte ferroviario che stradale. Mi permetto rapidamente di fare un piccolo elenco: mi riferisco alla riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno, al nuovo collegamento ferroviario transfrontaliere Arcisate-Stabio, alla tratta Arcisate-confine di Stato, al raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara, alla tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina, al potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno-Variante di Galliate, alla Variante di Galliate, per passare poi alla tangenziale ovest di Galliate, al collegamento diretto tra l'interconnessione RFO di Novara ovest e la linea FNME Novara-Malpensa, al potenziamento della linea Rho-Arona, alla tratta Rho-Gallarate, oltre - per concludere, l'elenco è lungo - all'indispensabile collegamento tra la Statale n. 11 «Padana Superiore» a Magenta e la tangenziale ovest di Milano, con la variante di Abbiategrasso e l'adeguamento in sede del tratto della strada statale n. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo Ponte sul Ticino. Mi avvio quindi a concludere sottolineando che non stiamo parlando solo di strutture, ma anche di persone, dei nostri lavoratori. È anche per loro che la Lega Nord si è sempre impegnata per il mantenimento dell'aeroporto di Malpensa.

io non penso che Malpensa sia un aeroporto padano, perché, se così fosse, la pratica sarebbe già chiusa e archiviata in quanto si tratterebbe di un problema della Regione Lombardia e della macroarea del Nord. Credo che il tema sollevato nelle mozioni presentate da tutti i Gruppi parlamentari sia qual è la politica del Governo rispetto al sistema aeroportuale italiano, quale il ruolo che questo ha nel contesto dei trasporti internazionali ed intercontinentali e come, dopo l'operazione Alitalia, si colloca nello scenario di questo sistema Malpensa, che non è più un *hub*,

noi l'abbiamo criticata fortemente - ma è una scelta che voi e questo Governo avete fatto e che determina oggi un ruolo diverso e certamente marginale di Malpensa rispetto a Fiumicino. Se noi dimentichiamo il passato, o riteniamo di occuparci di tali questioni in maniera occasionale e demagogica, questo Paese non andrà da nessuna parte. Il problema di Malpensa si pone partendo dal presupposto che, nonostante la scelta fatta dal Governo (giusta nel momento in cui si è trovato a dover scegliere dove organizzare il sistema sistema trasportistico di Alitalia e avendo scelto Fiumicino), il baricentro del sistema è diventato Fiumicino.

Sono stato derogate norme comunitarie e si è attivato un sistema di protezione sociale che non ha mai avuto eguali nel nostro Paese, anche sotto il profilo della tutela dei lavoratori. Tutto questo ha comportato una scelta che ha penalizzato e marginalizzato Malpensa. Nonostante ciò, poiché esistono consistenti fette di mercato, Malpensa ha vissuto vissuto ed è sopravvissuta, tanto è vero che i dati del bilancio della SEA fanno registrare un utile - come dichiara il suo Presidente - di 52 milioni di euro.

non dare per acquisito il dato di una scelta politica che l'Esecutivo ha fatto su questa materia, privilegiando il sistema Alitalia e Fiumicino. In questo contesto, è evidente che deve cambiare anche il sistema di governo In che senso? Essendo la società che lo gestisce partecipata, ad esempio, dal Comune di Milano ed essendoci degli utili, questi devono essere finalizzati

nazionale e internazionale di cui tutti dobbiamo farci carico e rispetto al quale c'è la necessità di una politica di sostegno a quel sistema dei trasporti in modo da agevolare la riuscita di un così grande evento. C'è poi l'esigenza di capire a che tipo di mercato ed a quale tipo di domanda deve assolvere Malpensa: il rischio qual è?

di sviluppo e rilancio di Malpensa, e quindi pensiamo di sostituire alla necessità di un piano strategico nazionale che riguarda tutto il sistema dei trasporti - in cui Malpensa ci sta perché i dati del mercato dicono che ci sta e ci sta bene e può starci ancora meglio e se tutto questo lo facciamo immaginando di intervenire con provvidenze su Malpensa per cercare di supplire ad una logica di mercato che è stata in qualche modo menomata dalla scelta fatta dall'Italia,

considerazione, affidando poi al dibattito e quindi all'intervento della collega Poli Bortone l'approfondimento di merito delle questioni. Credo che il punto centrale di cui dobbiamo discutere sia il seguente. In questi giorni alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale si sta discutendo di un provvedimento che riguarda il cosiddetto federalismo demaniale, cioè il trasferimento di una serie di beni dallo Stato

ci dice che cosa vuole fare del sistema aeroportuale italiano (se intende trasferirlo in tutto o in parte alle Regioni o agli enti locali o se invece ritiene che si debbano fare delle scelte strategiche, per cui vi sono degli aeroporti che hanno una loro funzione funzione nazionale e internazionale), e se non comprendiamo quali politiche si accompagnano a questo tipo di scelte evidentemente anche il dibattito di oggi rischia di essere un po'

da questo punto di vista forse il dibattito di oggi qualche passo avanti lo possa fare. Certamente, non considereremo un passo avanti l'idea che le mozioni approvate da questo ramo del Parlamento siano funzionali a qualche intervento assistenziale in più per qualche categoria che si trova scoperta rispetto alle scelte che il Governo ha fatto, perché, se fosse così, saremmo totalmente contrari.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi parliamo ancora una volta di Malpensa. Ricordo che due anni fa in quest'Aula ci furono degli accesi dibattiti, perché non si era capita l'importanza, a mio avviso,

nell'Italia del Nord e che difficilmente i nostri imprenditori con la valigetta, che vanno in tutto il mondo per vendere i nostri prodotti, avrebbero utilizzato l'*hub* di Roma, ma avrebbero privilegiato - ahimè, com'è successo

assolutamente necessario, dacché ci attendiamo oltre 20 milioni di visitatori, far sì che Malpensa ritorni ad essere un *hub* intercontinentale assolutamente sganciato dalla compagnia di bandiera, ma in ogni caso agganciato alle compagnie che hanno visto con estrema acutezza quello che Malpensa può rappresentare: un *hub* intercontinentale europeo.

e per l'Europa, produrre di concerto con le Regioni del Nord un *action plan* da cui si evincano i ruoli e le funzioni dei vari impianti aeroportuali gravitanti nelle rispettive Regioni, in modo da realizzare opportune sinergie anche in considerazione del modificato quadro dell'offerta di trasporto aereo. identificare un piano operativo che garantisca l'offerta organica delle infrastrutture legate all'accesso all'impianto aeroportuale che, com'è stato evidenziato, ha conosciuto dei grandissimi miglioramenti sotto il profilo della mobilità e della raggiungibilità di Malpensa. a sbloccare, quanto prima possibile, tutte le altre opere già approvate dal CIPE nella XIV Legislatura, direttamente o indirettamente collegate con l'aeroporto di Malpensa;

la mozione n. 275, presentata dal Gruppo dell'Italia dei Valori, è l'ennesimo tentativo di impegnare il Governo a dare piena attuazione agli impegni assunti negli anni sulle politiche di rilancio dello scalo di Malpensa sul potenziamento del sistema della mobilità, che non riguarda solo le grandi vie di accesso all'aeroporto, ma anche la rete complessiva che costituisce il supporto al sistema urbano. la necessità di prendere atto, una volta per tutte, di quel che è stato fatto e di quello che rimane ancora da fare per costruire un vero sistema aeroportuale in grado di competere a livello internazionale. L'indagine conoscitiva realizzata dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati sul sistema aeroportuale italiano delinea un sistema diffuso, ma debole e scarsamente idoneo a fronteggiare le potenzialità di crescita del traffico aereo, definito nello stesso documento conclusivo un sistema in difficoltà. Tale condizione dipende, in parte, da carenze ed inadeguatezze già rilevabili, come la scarsa accessibilità intermodale, causata dall'insufficienza dei collegamenti con la rete ferroviaria e stradale, e un livello di servizi in molti casi insoddisfacente. Il motivo di maggiore preoccupazione che emerge da tale indagine, tuttavia, non si riferisce tanto alla situazione attuale, ma a quella che si potrà determinare nei prossimi anni, e questo credo sia per noi È interesse generale e prioritario utilizzare le scarse risorse disponibili per ammodernare, ampliare e potenziare, in modo mirato, gli aeroporti già esistenti. In un tale contesto, l'aeroporto di Malpensa è il classico caso di scuola che diventa caso concreto. Mi piace ricordare l'*incipit* di un articolo del quotidiano «la Repubblica» del 10 marzo 2008 che, in piena crisi Alitalia, diceva: «Nessuna pietà per Malpensa». A distanza di due anni, si potrebbe riutilizzare sullo scalo lombardo la stessa identica espressione. Quello che potremmo definire il caso Malpensa si intreccia, com'è noto, con le travagliate e complesse vicende del caso Alitalia, con le vicende cioè di una compagnia per la quale, per anni, si sono unite gestioni irresponsabili a capitalizzazioni inutili. L'evoluzione del caso Malpensa si correla inevitabilmente, dunque, con le scelte riguardanti il salvataggio del vettore nazionale da parte di altri vettori, per certi aspetti interessati - come nel caso di Air France - ad investire proprio sullo scalo lombardo, sviluppandone le caratteristiche di *hub*, per lasciare, invece, all'aeroporto di Fiumicino il ruolo di scalo *point to point* destinato soprattutto alla clientela *business*. Siffatto orientamento verrà gradualmente invertito nella strategia di Air France-KLM che, in concorrenza con Lufthansa, relativamente alle vicende del progetto Fenice punterà alla valorizzazione di Fiumicino come scalo d'appoggio per le rotte verso l'Africa ed il Medio Oriente, con l'inevitabile e conseguente declassamento dello scalo di Malpensa. a distanza di più di dieci anni dalla sua inaugurazione come aeroporto intercontinentale, dopo due anni dalla conclusione della vicenda legata alla privatizzazione dell'ex compagnia di bandiera, il Governo non ha fatto molto per cercare soluzioni alternative alla non praticabilità del rilancio di Alitalia a Malpensa e ancor meno per il rilancio dell'intero sistema aeroportuale lombardo. Non si sono tenute in considerazione le potenzialità del sistema economico che gravita intorno allo scalo di Malpensa, nonostante - come è già stato evidenziato - il mondo imprenditoriale abbia manifestato a gran voce quanto lo sviluppo di Malpensa rappresenti per Milano e per la Lombardia una necessità imprescindibile per rafforzare le relazioni con tutti i principali mercati. Il nodo cruciale della questione dell'aeroporto di Malpensa è che esso soffre di un'accessibilità inadeguata, che ne fa troppo spesso una scelta secondaria per gli stessi viaggiatori dell'Italia nord-occidentale. Si sono succeduti negli anni interventi a livello comunitario, nazionale e regionale mirati a garantire l'offerta organica delle infrastrutture legate all'accesso all'impianto aeroportuale. Voglio brevemente passare in rassegna alcune delle misure adottate. Le strutture aeroportuali dello scalo lombardo sono state indicate come componenti di uno dei due unici impianti intercontinentali del Paese dal piano generale dei trasporti approvato nel maggio 1986, e sempre riconfermato nei successivi aggiornamenti; l'impianto aeroportuale intercontinentale di Malpensa è stato altresì considerato dal Consiglio europeo quale nodo aeroportuale chiave del sistema dei grandi *hub.* Nel 1994, il Consiglio europeo ha individuato un elenco di undici progetti prioritari nel settore dei trasporti, di cui tre riguardavano in modo diretto il nostro Paese, ed in particolare uno dei tre riguardava proprio Malpensa. L'inserimento dell'impianto aeroportuale lombardo all'interno di tale elenco ha comportato anche un adeguato supporto economico da parte dell'Unione europea. Durante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, nel 2003, è stato approvato il nuovo assetto delle reti TEN, al cui interno compaiono i tre corridoi plurimodali che interessavano direttamente il nostro Paese ed in particolare i tre corridoi al cui incrocio si trova Malpensa. Nella XIV legislatura il CIPE ha approvato un piano decennale delle infrastrutture strategiche al cui interno è stata prevista una serie di interventi legati al completamento delle opere stradali, ferroviarie e metropolitane di accesso all'impianto aeroportuale di Malpensa. Dal 2001, alcuni passi in avanti sono stati fatti con l'apertura il 31 marzo 2008 della superstrada Malpensa-Boffalora, il completamento del tunnel ferroviario di Castellanza e l'apertura dei cantieri della Pedemontana lombarda e della ferrovia Arcisate-Stabio; ma moltissimo resta ancora da fare - come si evince dal rapporto realizzato da Assolombarda, Confindustria Genova e Unione industriale di Torino presentato a febbraio 2010 a cominciare, soprattutto in vista dell'Expo 2015, dal potenziamento della tratta ferroviaria Rho-Gallarate prevista con delibera CIPE del 6 marzo 2009; dal raccordo tra Ferrovie Nord e Ferrovie dello Stato per far viaggiate i treni verso Malpensa indifferentemente sulle due linee; fino al collegamento ferroviario tra i Terminal 1 e 2 dello stesso aeroporto. aeroporto. Dopo aver tratteggiato questo quadro, in sostanza, quello che chiediamo nella nostra mozione è che il Governo si impegni, una volta per tutte, a superare le difficoltà poste in essere dall'attuale assetto normativo e regolamentare, mostratosi sino ad oggi incapace di gestire la complessità del sistema del trasporto aereo italiano, ed in particolare dello scalo di Malpensa, affinché vi sia una maggiore chiarezza dei ruoli e delle relazioni tra gli attori coinvolti a livello centrale e regionale. Il Governo deve adottare tutti gli strumenti possibili per razionalizzare l'uso delle attuali strutture e dare un servizio migliore ai cittadini utenti; deve impegnarsi a confermare il piano di investimenti per la realizzazione delle opere finalizzate a connettere in modo efficace l'aeroporto di Malpensa con il suo bacino d'utenza, nonché individuare nuovi collegamenti intercontinentali per il rilancio dell'intero sistema aeroportuale in questione, prestando la massima attenzione alla difesa dei livelli occupazionali esistenti, che per certi aspetti sono in pericolo. Il Governo si impegni dunque a costruire e a sviluppare un vero e proprio *network* in grado di produrre un'offerta commerciale competitiva con i grandi aeroporti del Centro-Nord, garantendo non da ultimo il rispetto dei territori coinvolti. Onorevoli colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Guglielmo Marconi» di Rovereto, in provincia di Trento, ai quali diamo il benvenuto.

la questione riguardante Malpensa, scorta da una certa angolazione, mi ha fatto tornare in mente un fortunato libro di Andrea Camilleri intitolato: «Il birraio di Preston». Qual è, in particolare, la specificità di questo libro? Ve la faccio breve: giunti all'ultima pagina, ci si rende conto che, mutando l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Ognuno dei diciotto capitoli di cui è composto esaurisce la storia, pur aggiungendo un particolare in più, cosicché il lettore si trova dinanzi ad un romanzo scritto a chiave, che teoricamente si può cominciare non necessariamente dal principio ma da qualsiasi punto. Voglio dire che, anche a prescindere da proiezioni, tabelle e numeri, il dato di fondo è che Malpensa - pur nell'accidentato cammino che l'ha vista protagonista rispetto alla vicenda della compagnia di bandiera - rimane e deve rimanere una grande opportunità, specie se considerata alla luce degli investimenti previsti per Expo del 2015. ormai consuetudine consolidata far risalire talune criticità e il lento volgere su un piano inclinato, con il consapevole disegno di voler fare di Malpensa la classica cattedrale nel deserto, soprattutto agli effetti

al di là dei proclami - nelle infrastrutture, o perché mai qualsiasi progetto di ampio respiro -l'ultimo esempio, senza entrare nei contenuti, sono le dichiarazioni sul nucleare - venga datato a partire dal 2013, cioè dalla fine prevista della legislatura. Credo, viceversa, che vi siano questioni riguardanti il bene del Paese sulle quali è giusto ed opportuno trovare consenso e - dal mio punto di vista - finanche convergenze fra l'Esecutivo e l'opposizione. Sarebbe infatti miope considerare Malpensa alla stregua di una problematica meramente regionale, collegata cioè al perimetro condominiale lombardo e posta in relazione esclusivamente agli snodi limitrofi di Linate, Orio al Serio e Brescia Montichiari. Va messo in campo non un discorso di parte, perché non siamo in presenza di un mero interesse settentrionale che ci si limita di fatto a sventolare come una clava per denunciare le inadempienze dell'Esecutivo, del quale poi paradossalmente qualcuno degli sbandieratori è parte integralmente. Valorizzare Malpensa, la sua forza lavoro e le sue enormi potenzialità, significa qualificare non solo un'area nevralgica e centrale della piccola e media impresa e dei suoi occupati, ma il Paese nel suo insieme. che si ha sotto i piedi e spingere avanti la prospettiva: vincere, insomma, la sensazione che si ha dinanzi a qualsiasi discorso concernente servizi e infrastrutture che, per annunciare una novità, implicitamente ci si debba ridurre a denunciare un ritardo. Ed è quanto mai sconveniente perseverare entro un paradigma che affronta solo in parte e nulla risolve, com'è quello della sterile e vuota contrapposizione tra Roma e Milano. Credo sia venuto il momento di passare dalle intenzioni ai fatti: promuovere, senza ulteriormente rimandare, una serie di misure che possano garantire continuità di crescita e fruibilità dei servizi, partendo dai collegamenti con lo scalo aeroportuale che sono fondamentali e oggi largamente largamente insufficienti. I dati di consolidamento oggettivi e di ripresa di Malpensa devono far riflettere e mi chiedo quanto sarebbe sciocco - questo vale anche per noi dell'opposizione sabotare il timone dopo aver così faticosamente rialzato le vele, in attesa che soffi il vento. Per questo ogni capitolo, ogni aspetto riguardante lo scalo milanese e il suo sviluppo, non può esaurirsi fra fastidio e fascino, resistenza e resa: da qualsiasi punto ci volgiamo per affrontare il problema, ne emerge la sua centralità non non periferica, lungo una deriva che oltrepassa con disinvoltura i confini platonici e rassicuranti di una inesistente Padania, per imporsi entro una cornice di ben altro respiro e più ampia per il bene del Paese.

che anch'io considero essere non certamente padano, ossia un aeroporto di una sorta di zona virtuale alla quale si fa riferimento troppo frequentemente nel nostro Parlamento. Intervengo piuttosto a difesa di un aeroporto italiano che oggi non riveste più quel ruolo importante che lo stesso I Governo Berlusconi del 1994 aveva voluto ritagliare in termini di strategicità

e, quindi, un punto di riferimento nazionale per i trasporti internazionali. Questa doveva essere la funzione di Malpensa. Ma credo che la vicenda Malpensa oggi paghi anche lo scotto di due problemi importanti: in primo luogo, la politica decisamente assistenzialistica - questa volta sì,

(che continua a mantenere una sorta di regime di monopolio, contribuendo con questo anche ad una forte discriminazione territoriale rispetto ai territori del Mezzogiorno d'Italia, che si trovano decisamente in uno stato di di sofferenza per la mancanza di libertà rispetto al sistema dei trasporti e quindi di collegamento, all'interno della nostra Nazione);

rivesta veramente quel ruolo di aeroporto italiano, con tutte le funzioni che competono ad un aeroporto di

In qualsiasi altra parte del mondo esistono piccole compagnie aeree che consentono trasporti del genere e che finiscono con il creare una parità di opportunità tra territori che dovrebbe essere alla base del federalismo;

percorrere la strada indicata dal collega D'Alia, che è quella del primo decreto attuativo sul federalismo, quello del federalismo demaniale,

per gli oneri, gli eventuali ricavi o, naturalmente, le eventuali perdite. Così non è e non deve essere rispetto ad un aeroporto che deve rivestire una funzione di livello nazionale

importantissima. Probabilmente si dovrebbe fare una politica di maggior raccordo, a livello nazionale, con Lufthansa. È pregevole il fatto che Lufthansa abbia disposto, se ricordo bene, nove voli che collegano, tra l'altro, anche la mia Bari, ma mi pare pochino come tipo di intervento per la garanzia di trasporti all'interno della nostra Nazione. Anche noi riteniamo peraltro che su Malpensa si debba intervenire in maniera massiccia e con una volontà unanime da parte quest'Aula anche in rapporto a quello che potrà essere Expo 2015.

di interventi, anche di carattere infrastrutturale, quale quello che stiamo sollecitando per l'aeroporto di Malpensa, ma anche l'occasione affinché l'intero territorio nazionale possa vivere di tutti quanti gli eventi collegati alla manifestazione, e quindi si possano creare le condizioni perché ciascuno di noi possa efficacemente partecipare.

purché sia vissuto in termini nazionali e internazionali. In questo senso siamo assolutamente a favore di tutti quanti quegli interventi che vorranno garantire questo tipo di funzione; una funzione che dovrebbe essere ben definita anche in tema di federalismo demaniale, e non solo,

che un aeroporto, per quanto collocato fisicamente nel Nord, rappresenti un momento importante di collegamenti, non soltanto fisici, ma anche di altro livello, rispetto all'intera Nazione e, in particolare, rispetto quei territori del Mezzogiorno d'Italia che ci stanno particolarmente a cuore e che vorremmo fossero coinvolti in qualsiasi tipo di attività e di risorse finanziarie cui il Governo finanziarie cui il Governo si senta fortemente impegnato, con il supporto - mi auguro - dell'intero Parlamento, ma soltanto con questo spirito nazionale. *(Applausi *(PD)*. Signora Presidente, intervengo molto brevemente a sostegno della mozione che ho sottoscritto e che ha ben illustrato il senatore Vimercati.

non è cambiato nulla rispetto agli impegni presi dal Governo nel 2008: nulla è stato fatto, in questi due anni, per Malpensa, anzi. Voglio dire di più: la nuova Alitalia, quella dei capitani coraggiosi, quella invocata per Malpensa e Linate, tanto sostenuta ad esempio dal sindaco di Milano Moratti e dal presidente della Lombardia Formigoni, quella che ci è costata, come ricordava il collega Vimercati,

dati alla mano, è andato tutto molto peggio, sia per gli aeroporti milanesi sia per quelli lombardi. La SEA, la società

lo spostamento verso le compagnie *low cost* (peraltro in concorrenza con gli altri aeroporti lombardi) la allontana e non la avvicina alla prospettiva di un grande aeroporto internazionale.

responsabilità, non si può certo sottacere l'inerzia anche delle grandi istituzioni locali: grande inerzia sia sul piano degli impegni concreti che nell'iniziativa politico-istituzionale nei confronti

Il tema dell'accessibilità di Malpensa è ormai drammatico e mette in forse l'attuazione dello stesso progetto di Expo 2015. Lombardia non ha fatto nulla sulla programmazione e sul coordinamento tra gli aeroporti lombardi; il Comune di Milano, da parte sua, legando tutto all'Expo, non ha dato priorità a Malpensa e alla sua accessibilità, con il risultato paradossale che non c'è ancora un cantiere avviato e che anche le risorse sono in forse. In compenso, il Comune di Milano, ha

Però, pensare di risolvere i problemi del bilancio in questa maniera è davvero inaccettabile. Concludo, signora Presidente, parlando appunto del

Di conseguenza, come si intende affrontare la drammatica situazione occupazionale che, come ricordato dai precedenti interventi, coinvolge circa 50.000 posti di lavoro? A queste domande il Governo deve assolutamente rispondere. Finora, Malpensa e i suoi lavoratori sono stati abbandonati al loro destino. È arrivato il momento di mantenere gli impegni presi.

intervenire alla conclusione di un dibattito consente di sfoltire il proprio intervento, perché moltissime considerazioni, in particolare quelle fatte ora dal collega Roilo, sono assolutamente condivisibili. Tenterò, quindi, una sorta di sintesi per fare una riflessione insieme a voi. Le mozioni che stiamo discutendo pongono in evidenza chiaramente come l'assenza di un piano nazionale dei trasporti e, in particolare, la mancanza di un piano di coordinamento, di razionalizzazione e di specializzazione delle infrastrutture, rendano il mercato Italia, soprattutto al Nord, più fragile e permeabile. Permeabile, per esempio, all'ingresso dei vettori *low cost*, che sono stati qui citati. Nessuno vuole demonizzare questo tipo di vettori, però questi, se da un lato contribuiscono ad aumentare l'offerta di accessibilità in termini di collegamenti punto a punto, dall'altro impediscono al sistema aeroportuale di potersi confrontare con un modello di sviluppo sostenibile nel medio e lungo periodo. Infatti, la mancanza di specializzazione produttiva e di differenziazione qualitativa dell'offerta dei passeggeri, unitamente a processi competitivi basati unicamente sul fattore prezzo, ha disincentivato gli investimenti in infrastrutture, depauperando negli anni la qualità complessiva del servizio e aumentando la conflittualità tra sistemi aeroportuali. Tale situazione, inoltre, ha prodotto un aumento del potere contrattuale da parte di alcune tipologie di operatori aerei e reso distorsivo e poco trasparente il sistema tariffario. Veniamo di nuovo a Malpensa. Un punto essenziale che è venuto fuori da diversi interventi è l'efficacia e l'efficienza del sistema Malpensa e la sua appetibilità per gli operatori. È opinione comune a tutti gli operatori che l'aeroporto di Malpensa potrebbe svolgere un ruolo maggiormente significativo per lo sviluppo economico del Nord se la sua accessibilità, in particolare per quanto riguarda la rete stradale e ferroviaria, fosse più efficiente. È, inoltre, altrettanto condivisa tra gli operatori del settore l'opinione che il programma di sviluppo di Malpensa risulterebbe più convincente se non vedesse coinvolte istituzioni pubbliche, alcune anche azioniste di riferimento (come ha appena ricordato il senatore Roilo), con interesse a drenare gli utili di gestione piuttosto che a investire. Istituzioni pubbliche e società private, compagnie aeree e società che erogano servizi a terra, hanno in molti casi difficoltà a condividere gli stessi obiettivi strategici e a conseguire un'efficace livello di integrazione. Il piano di investimenti presentato da SEA al Governo il 14 ottobre 2009, stando anche ai risultati presentati ieri, sembra dare i primi frutti, ma questo non basta. Ad esempio, va decisamente troppo a rilento la preannunciata rinegoziazione dei diritti di volo che potrebbe aprire nuove e importanti opportunità di *business* proprio per l'aeroporto di Malpensa. Malpensa. Per sintetizzare il nostro punto di vista sull'argomento si può sostenere che, oltre a tempi e risorse compatibili con i *trend* di sviluppo del mercato, è necessario condividere un approccio metodologico i cui elementi imprescindibili non possono che essere i seguenti: pianificazione puntuale e preventiva dello sviluppo delle infrastrutture aeroportuali; miglioramento dell'accessibilità con particolare riferimento ai collegamenti con l'alta velocità e l'alta capacità ferroviaria; forte incremento dell'intermodalità; definizione di livelli minimi di servizio correlati alla qualità di strutture e infrastrutture in termini di funzionalità e *comfort* per gli utenti; contenimento di consumi energetici; relazione con l'ambiente e il paesaggio. Solo se la qualità del servizio e la sostenibilità economica rappresenteranno l'obiettivo comune di tutti gli operatori della filiera del trasporto aereo, l'aeroporto di Malpensa potrà rappresentare quel volano di sviluppo economico che tutti qui hanno auspicato. la chiusura di fatto dell'*hub* di Malpensa è stata sicuramente molto negativa, perché ha fatto quasi cessare gli impatti tipici di un grande *hub* intercontinentale. L'impatto diretto è evidente; l'impatto indiretto è meno evidente, ma in crescita: non dimentichiamo che le attività cosiddette *non aviation* rappresentano oggi circa la metà dei ricavi delle gestioni aeroportuali negli aeroporti europei.

delle imprese *high tech* e per quanto riguarda la catena logistica delle merci ad alto valore che sono molto importanti per il sistema produttivo italiano. Ma al tempo stesso la situazione che si è determinata è una contingenza storica molto strana e potenzialmente molto favorevole: si ha, come riconosciuto da molte mozioni, un eccesso di offerta di infrastruttura e, nello stesso territorio, un eccesso di domanda di servizio di trasporto aereo. si crea nel mercato un vuoto, che il mercato tende a riempire, e tende a riempirlo soprattutto in capo a quei soggetti che esprimono contemporaneamente una forte domanda di infrastruttura e l'offerta del servizio aereo, cioè le compagnie aeree. Allora, nel condividere molto di quanto detto dalle mozioni, vorrei tuttavia segnalare un aspetto, e cioè che molto della rendita propria del *business* aeroportuale rischia oggi di

italiano. Attenzione: non sono preoccupato dal fatto che Malpensa resti un aeroporto vuoto per molti anni: si riempirà, ma si riempirà di collegamenti internazionali operati da compagnie straniere, come sta già avvenendo,

dal fenomeno delle *low cost*, ma non solo: si sono effettivamente ridotte tutte le barriere che proteggevano le compagnie aeree tradizionali e che oggi rendono la scelta dell'operatore, del vettore aereo, rispetto all'infrastruttura aeroportuale molto più volatile. Questo è un grande rischio non basta più investire e non è più così facile investire, perché l'investimento ha un rischio molto maggiore di quanto non avesse prima. Partendo da queste considerazioni, vorrei più che altro sottolineare che molti degli intendimenti previsti dalle mozioni, in particolare da quella a prima firma del senatore Butti, sono sicuramente condivisibili. Rammento, in particolare, quello che è stato ricordato anche nell'intervento che mi ha preceduto, di individuare ruoli e funzioni del sistema

dell'accessibilità terrestre all'aeroporto, su cui sono necessari maggiori investimenti. Tuttavia, certamente vanno ricordati altri aspetti; il primo è quello delle liberalizzazioni vere ed effettive: mantenere monopoli in capo al trasporto aereo e agli aeroporti oggi in Italia ha Attenzione: non è che vi sia troppo poca protezione su Malpensa, ce n'è troppa su Fiumicino e sull'Alitalia. Dobbiamo favorire maggiori liberalizzazioni, affinché la rendita del *business* aeroportuale non venga catturata da operatori che nulla hanno a che fare con l'economia italiana. Da questo punto di vista, sarebbe anche importante sprovincializzare la gestione dell'aeroporto, fondamentalmente in due modi: attirando compagnie straniere nelle compagini azionarie e quindi cercando di legarle al rischio dell'investimento su Malpensa e cercando partner industriali sulla gestione aeroportuale che siano grandi gruppi internazionali, e non solo società italiane.

negli anni scorsi, si è parlato molto ed ora possiamo anche aggiungere, senza ipocrisia, che spesso si è parlato a sproposito, in qualche caso senza conoscere in profondità le questioni. Ho riletto i resoconti stenografici di diverse sedute tenutesi negli ultimi due anni e mi sono anche un po' divertito, devo ammettere, perché sono stati evocati disastri e catastrofi; la rassegna stampa portava pagine di apocalissi, che puntualmente poi non si sono verificate. Ricordo servizi giornalistici che rappresentavano la condizione di Malpensa abbandonata dalla compagnia di bandiera come irreversibile, cosa che poi abbiamo dimostrato non essere. Forse, colleghi, era proprio Alitalia il problema di Malpensa, e non il contrario! Certo, l'abbandono di Malpensa da parte di Alitalia ha prodotto guasti di notevole entità, sotto il profilo sociale, occupazionale e sotto il profilo economico in buona parte della Lombardia ma non solo. Ma il Popolo della Libertà era ottimista, e non perché avesse un debole per le favole a lieto fine, bensì perché aveva valutato diversamente dai colleghi del centrosinistra le opportunità che si stavano prospettando per il rilancio di Malpensa. In effetti, basta leggere anche i giornali di oggi per vedere che vi è stato un prodigioso recupero, sia per il passaggio delle merci, sia per il transito dei passeggeri; e se a questo si aggiunge il ritorno di ben 185 voli internazionali possiamo ben dire che Malpensa stia risalendo la china. Sia chiaro, non siamo evidentemente ancora soddisfatti, ma confermiamo l'ottimismo: Malpensa produce utili. Quello stesso ottimismo che anche durante il ridicolo, paradossale *derby* con Fiumicino non abbiamo mai smarrito perché sapevamo e sappiamo perfettamente - i dati ci danno ragione che Malpensa e Fiumicino potevano essere realtà, se non addirittura complementari come poi si è dimostrato, comunque in grado di vivere autonomamente all'interno di un disegno nazionale, organico, per il trasporto aereo. E così è stato. Ricordo anche le fantasie sulle chiusure del *city airport* di Linate: lo ricordiamo tutti quanti. Oggi l'Italia, la Lombardia, Milano e quindi Malpensa si affacciano alla frenetica organizzazione dell'Expo 2015 con la serenità che deriva da due certezze: della prima - la certezza offerta dal Governo nazionale con il suo piano infrastrutturale, che sta procedendo, nonostante le Cassandre, ad ampie falcate, nonostante la crisi economica E la seconda certezza è la grande forza produttiva della Lombardia che, come è stato riconosciuto e ricordato, produce un PIL quasi simile a quello di uno Stato sovrano come l'Olanda. che tutti gli attori protagonisti nei vari livelli istituzionali, Regione Lombardia compresa, stanno esercitando per valorizzare Malpensa quale strategico crocevia tra il Corridoio dei mari Rotterdam-Genova, tra il Corridoio Lisbona-Kiev e Berlino-Palermo, non non possiamo far altro che esprimere buoni auspici rispetto alle previsioni di crescita del trasporto aereo passeggeri del Nord Italia, che passerà dai 49 milioni del 2004 a 101 milioni del 2021. Una grande, grandissima, straordinaria opportunità. La nostra mozione, illustrata dal presidente Cantoni, serve a fare il punto della situazione per portare a conoscenza - certamente del Parlamento, ma anche dell'opinione pubblica - le politiche in atto per il rilancio di Malpensa: politiche che sono in continua e costante evoluzione per il contributo di tutti. E noi che dal nostro osservatorio privilegiato, che è l'8a Commissione Senato, conosciamo il cronoprogramma delle opere previste per l'Expo 2015, abbiamo la necessità di capire quando le altre opere, già approvate dal CIPE, vice ministro Castelli, e in quale modo verranno poi collegate allo sviluppo di Malpensa. E sappiamo anche del grande lavoro svolto dal Governo circa le politiche europee di *Open Skies*, politiche che sicuramente vedranno Malpensa protagonista. Però abbiamo l'esigenza - mi avvio alla conclusione - di sentire anche altro. In ordine ad esempio alla realizzazione della terza pista, per la quale il Ministero della difesa ha già ceduto il terreno necessario, o alla revisione dei trattati bilaterali extra Unione europea in vigore tra l'Italia e gli altri Paesi per consentitemi di utilizzare un termine forse non del tutto adeguato - liberalizzare l'operatività di tutti i vettori. In conclusione, Presidente, il sistema produttivo lombardo e quindi il sistema produttivo italiano ha, come noi del Popolo della Libertà, una grande fiducia nel futuro di Malpensa: una fiducia che riteniamo essere riposta nel modo migliore.

Grazie dei punti assolutamente condivisibili: da un lato, la sincera volontà da parte di tutti di promuovere lo sviluppo di Malpensa, considerato come uno dei punti di forza del sistema aeroportuale italiano, e dall'altro una serie di proposizioni nei dispositivi delle mozioni che sono in larghissima parte condivisibili perché, appunto, propongono una serie di azioni volte a continuare a sviluppare questo importantissimo aeroporto. C'è un punto molto delicato su cui vorrei attirare l'attenzione dei colleghi e rispetto al quale in questo momento il Governo propone delle modificazioni ai dispositivi delle mozioni. Intanto vorrei dire questo: colgo in molti interventi, peraltro fatti in assoluta buona fede,

Se ciò era positivo dal lato dell'erogazione del servizio, si è rivelato disastroso per le casse dello Stato. Ricordo che le Poste macinavano pesantissimi passivi;

compagnia aerea - la vicenda è nota - era oberata da un numero enorme di dipendenti, con conseguenti costi, e macinava grandi passivi. L'aspetto positivo, forse, era che il Parlamento e il Governo potevano intervenire in maniera massiccia sulle scelte strategiche e di trasporto di questi sistemi, cercando di adeguarle alle esigenze

ci troviamo di fronte agli stessi vettori, che però, a seconda degli scali che utilizzano, devono sottostare a diverse regole. All'interno del nostro Paese e dell'Europa, dobbiamo sottostare alle regole della Comunità europea, e quindi siamo in un sistema che è liberalizzato. A livello internazionale dobbiamo invece sottostare ad un sistema che è ancora completamento dirigistico, dirigistico, per il quale occorre evidentemente sviluppare accordi bilaterali, e quindi non c'è alcuna facoltà da parte degli operatori di agire in piena libertà. di un altro cambio di scenario, al contrario di quanto accade in questo momento in alcuni importanti mercati, come gli Stati Uniti, dove invece opera Skies*. Per complicare ancora di più il quadro, sappiamo che in questo momento, soprattutto per gli accordi bilaterali, la Comunità europea raccomanda accordi non tra Stato e Stato, ma tra Stati e Comunità europea: questo va a complicare vieppiù il quadro. ormai calarci in tale situazione, altrimenti non si potrebbe capire cosa il Governo può fare e cosa non può fare. E qui entro nel punto delicato di moltissime mozioni:

Il Ministero delle infrastrutture e l'ENAC hanno finanziato uno studio sullo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali che è ormai in fase di stesura definitiva. Tale studio è volto a costruire una fotografia dell'attuale contesto, redatta in maniera omogenea per tutti gli aeroporti, al fine di facilitare la lettura e la trattazione dei dati. Su tale base viene poi esaminata e valutata l'interazione con il territorio e con le altre modalità di trasporto. Sono considerati i contesti socio-economici, la capacità attrattiva, la capacità turistica della zona in cui gli aeroporti si trovano. Infine, vengono esposte le criticità che il sistema aeroportuale presenta, al fine di consentire valutazioni appropriate. Tanto premesso, rimane però alle compagnie aeree la scelta delle opportunità offerte operando concretamente i voli, senza possibilità di condizionamenti da parte delle autorità,

Sta realizzando uno studio, che poi metterà a disposizione delle compagnie aeree e ovviamente delle società di gestione degli aeroporti, per porre in essere un'azione di natura persuasiva affinché le compagnie aeree possano scegliere le opportunità che meglio credono. Questo è quanto al massimo possiamo fare: quindi,

Voglio dire che, non è che avendo sottoscritto un accordo bilaterale, poi automaticamente abbiamo il servizio, perché potrebbe tranquillamente darsi che un certo tipo di collegamento che il Governo sottoscrive con l'omologo Stato non venga ritenuto appetibile da nessuna compagnia. Su questo punto, cosa abbiamo fatto per Malpensa?

che accusano questo Governo di essere stato in parte causa della crisi di Malpensa: badate, colleghi, che il *de-hubbing* di Malpensa è avvenuto a marzo del 2008, quando la compagnia Alitalia era di piena di piena proprietà del Governo, e il Governo non era certamente il nostro. La crisi di Malpensa nasce da quel giorno: in quel momento Malpensa perde di colpo quasi 10 milioni di passeggeri. La susseguente scelta di Alitalia di assumere come *hub* principale Fiumicino e non Malpensa avviene - è vero - sotto il Governo Berlusconi, ma in un contesto completamente cambiato, perché in quel momento Alitalia diventa una compagnia pienamente privata che opera seconda logiche private. È del tutto noto che una parte importante

*hub* italiano per quanto riguarda il trasporto delle merci. Poi finiamola, per cortesia, di dire che Malpensa è un deserto. Malpensa, malgrado il *de-hubbing* che ha provocato i noti risultati, ha portato l'anno scorso 18 milioni di passeggeri. Mi domando come si fa a definire deserto il secondo aeroporto italiano che, insieme a quello di Linate - che è poi di fatto il sistema aeroportuale milanese - vede trasportare 28 milioni di passeggeri, con un *trend* di crescita che, lo ripeto, è in controtendenza rispetto a tutta l'Europa e a tutto il mondo. Si tratta di dati incontrovertibili ed incontestabili,

Ebbene, anche da questo punto di vista, possiamo però dire con orgoglio che non è stato licenziato neanche un lavoratore dalla SEA,

in maniera ottimale, non essendo stato licenziato neppure un lavoratore, e ciò non è testimoniato soltanto dalle mie parole, ma dal fatto molto più importante che, in tale contesto, i lavoratori della SEA non hanno fatto neanche un'ora di sciopero, e tutto è avvenuto in perfetto accordo

signori, c'è un punto su cui bisogna mettersi d'accordo. È chiaro che l'infrastrutturazione dei sistemi di trasporto che portano verso Malpensa si colloca sostanzialmente all'interno

della stampa e dell'opposizione che non facciamo niente, mentre poi puntualmente al CIPE vengono finanziate le opere e vengono aperti i cantieri, e questo accade in continuazione.

consentirà di portare a Malpensa tutto il bacino del Canton Ticino, che è economicamente molto interessante.

in previsione, opere progettate e cantierate, stiamo parlando già di più di un miliardo di investimenti. Questo è dunque il quadro oggettivo della situazione

al punto in cui l'Esecutivo viene invitato, in un modo più o meno dirigistico, ad intervenire sul contesto della specializzazione dei vari aeroporti. Questo, però, non si può fare. Allora, entrando nel merito,

Grazie

non possiamo abolire queste tariffe. Ricordo che i piani di infrastrutturazione all'interno degli aeroporti, predisposti dalle società di gestione e, quindi, in maniera virtuosa e senza gravare sulle tasche dei cittadini italiani, vengono realizzati proprio con gli introiti delle tariffe. Ricordo altresì che le nostre tariffe, ed in particolare quelle di Malpensa, sono del 35 per cento inferiori rispetto alla media europea.

rispetto alla considerazione delle funzioni di un aeroporto che attualmente non sono ancora ben definite, ma comunque investono l'attenzione di tutto il territorio nazionale, e non soltanto di un territorio. Ci è sembrato, invece, che il ministro Castelli volesse ricondurre in una sorta di recinto geografico un problema che noi intendiamo affrontare a livello di problema nazionale.

diminuzione dei costi e quindi delle diverse tariffe dei vari servizi pubblici, il fatto di non accedere ad una richiesta del genere in un momento di forte crisi quale quella che sta attraversando l'Italia

Sinceramente non comprendiamo il motivo per il quale dovremmo rimodellare questo nostro suggerimento e soprattutto la nostra linea di indirizzo. Il mettere mano ad un piano aeroportuale italiano significa, soprattutto in termini di politica generale dei trasporti, cercare di mettere ordine in un sistema che effettivamente oggi non funziona.

commettendo - secondo me - una imprecisione, là dove ha attribuito al Governo Prodi la responsabilità iniziale del *default*

Dopo essere stato un campo di volo militare, durante l'ultimo conflitto venne

le basi per poi creare un grande aeroporto per tutto il Nord

rivedere un po' la situazione del rilascio degli *slot* per preservare al sistema aeroportuale milanese quelle caratteristiche e potenzialità che può avere. Dobbiamo plaudire anche a SEA, nella persona del suo presidente, che pure in una situazione di recessione economica è riuscito a mantenere i bilanci non in rosso.

e anche per questo proverò a rendere l'intervento più breve, salvo dire al senatore Leoni che

La discussione ci è apparsa per alcuni versi fuori contesto, per altri fuori tempo, per altri ancora fuori dalle nuove normative che, fra l'altro, anche il Vice Ministro ha richiamato. D'altronde le mozioni le abbiamo lette. Tutte impegnano il Governo a negoziare o rinegoziare i diritti di volo con i Paesi esteri interessati, alcune dimenticando che in parte si tratta di una norma già approvata dal nostro Parlamento, altre non considerando affatto il ruolo dell'Europa. Quasi tutte le mozioni auspicano una sorta di piano aeroportuale del Nord, declinandolo in vario modo: «piano di coordinamento», «piattaforma di coordinamento», «piano di azioni». Tutte le mozioni si richiamano all'Expo 2015 e alle opere di collegamento con l'aeroporto. Infine, giusto non farci mancare nulla, in tutte le mozioni si fa riferimento alla crisi occupazionale dell'area. L'incremento L'incremento di traffico aereo registrato nel decennio passato e, soprattutto, l'incremento previsto per il prossimo decennio impongono un ragionamento non più differibile di riorganizzazione nazionale che sappia però tener presente la progressiva liberalizzazione del traffico aereo dovuta alla normativa comunitaria. Molti interventi che ho ascoltato non guardano al cliente finale, non guardano ai vantaggi della liberalizzazione; anzi - alla faccia della liberalizzazione! - in nome delle risorse già impegnate si chiede in fondo di tutelare e di difendere l'esistente,

a una discussione sul trasporto aereo nazionale. Immagino ci saranno linee guida, criteri oggettivi, strategie di investimento, ipotesi di sviluppo che riguardano l'intero sistema Paese. Ma possiamo veramente essere interessati a discutere della questione Malpensa come se si trattasse di un piano delle Province di Milano, Varese e Brescia?

Ma perché non presentare allora una mozione che riguardi l'Expo? Perché fermarsi solo su Malpensa? O su ogni opera che riguarda l'Expo dovremmo fermare il Senato a discutere di mozioni specifiche? Alla fine, l'unico impegno che sembra rimanere concreto e sostanzioso è quello che vorrebbe estendere i benefici previsti per gli ex lavoratori Alitalia a tutti quelli dello scalo, e addirittura ai lavoratori dell'indotto. Si trattasse di altre parti del Paese, si parlerebbe di assistenzialismo. Purtroppo è di ieri la notizia che la società di gestione di Malpensa realizza utili.

a tutte quelle mozioni che trattano Malpensa come uno scalo regionale, come uno scalo lombardo. Quelle mozioni, e chi le ha scritte, declassano l'aeroporto di Malpensa, non considerandolo scalo nazionale indispensabile allo sviluppo di tutto il Paese. I piani

noi guarderemo con grande attenzione alle mozioni che vogliono Malpensa scalo nazionale ed internazionale di grande valore, e non a quelle che considerano Malpensa come un piccolo aeroporto di due o tre Province del Nord Italia.

il merito di questa mozione, voglio sottolinearlo anch'io, è quello non solo di aver mantenuto, praticamente intatta, la sua validità e attualità, ma anche di consentirci di guardare, ormai con sufficiente distanza temporale e adeguato distacco emotivo a che cosa si è consumato con la vicenda Alitalia; a che cosa non è stato colto, non solo dall'opinione pubblica, ma anche nel nostro dibattito politico, nonostante, o forse proprio a causa, della sovraesposizione mediatica registrata in quei mesi, che coincisero, voglio ricordarlo, con la fine infausta di una legislatura e con la celebrazione, forse prematura, dei fasti di quella nuova, l'attuale, che proprio a partire da quella vicenda ha probabilmente innovato uno stile di Governo, tanto nella comunicazione, quanto nelle procedure parlamentari, quanto nell'azione di Governo stessa. Uno stile che ha drammaticamente coinciso con un'alterazione della sostanza dei fatti dalla realtà effettiva delle cose. Anche in questa vicenda sì è assistito infatti al rilievo, direi abbagliante, che è stato conferito ad alcune questioni e, contestualmente, al precipitare in un cono d'ombra di altre. Fu infatti attribuito alle sorti della compagnia Alitalia il valore di *asset* strategico per il sistema Paese, ma non altrettanto fu considerato, alla stessa e maggiore stregua il sistema degli scali aeroportuali o la quantità e la qualità dei collegamenti effettivi del nostro Paese, da e verso il resto del mondo, che già allora avrebbero dovuto vedere una gestione più dinamica degli *slot*, come del resto prevede un mercato liberalizzato. La vicenda Malpensa ha in sé questa cifra e noi oggi ve la riproponiamo pressoché identica. Da rilevare in positivo, da allora, l'intraprendenza della società di gestione dello scalo aeroportuale che ci consente di apprezzare, non certo la sensibilità del Governo, che ha congelato finché ha potuto gli *slot* non utilizzati da Alitalia, ma la vitalità di quel tessuto dell'economia italiana, che ha scongiurato il naturale declino che sarebbe dovuto conseguire dal *de-hubbing* di Alitalia, un evento che ha comportato - come è stato ricordato - la perdita di 10 milioni di passeggeri. Oggi - veniva ricordato - a distanza di due anni, segnali confortanti di ripresa, pur non registrandosi ancora, è bene sottolinearlo, nel numero dei passeggeri, che costituiscono l'indicatore principale di salute di uno scalo, sono costituiti dalla sostituzione degli *slot* inutilizzati con nuovi voli, che hanno riportato ad un complessivo di 160 destinazioni rispetto alle precedenti 166, di quando Alitalia costituiva l'80 per cento del complessivo. Probabilmente l'esperienza consumata ci induce a ritenere, come rileva, a mio avviso giustamente, anche l'indagine conoscitiva richiamata, promossa dai colleghi della Camera, che una gestione più dinamica delle tracce orarie (gli *slot*) è la risorsa principale di uno scalo e di conseguenza occorre che il Governo avvii un profondo ripensamento sul ruolo improprio che ha fatto giocare ad ENAC in tutta questa vicenda. La riforma di un nuovo sistema di «*governance*» del trasporto aereo costituisce una priorità non oltre procrastinabile. Ma il punto centrale della questione, che la mozione n. 11 (testo 2) presentata dal senatore Vimercati evidenzia, è la dotazione infrastrutturale di collegamento degli aeroporti alle principali arterie ferroviarie e autostradali, come puntualmente è stato indicato appunto nella mozione che abbiamo presentato e che per questo non riprendo nel dettaglio. questione particolarmente avvertita per Malpensa, ma purtroppo condizione diffusa per la maggioranza dei nostri scali portuali e aeroportuali, come evidenziano i molteplici studi di settore che richiamava anche il Vice Ministro. È questa per noi la priorità delle priorità infrastrutturali per il nostro Paese, non avvertita ancora, purtroppo, nell'azione di questo Governo. La situazione vede le nostre porte di accesso naturali per merci e per passeggeri o congestionate nel contesto urbano o più spesso purtroppo relegate in contesti isolati e non collegati adeguatamente dal punto di vista infrastrutturale. Proprio questa è stata ed è tuttora la principale causa del mancato sviluppo atteso per Malpensa e di converso la principale ragione del prolificare di una serie di scali ravvicinati che hanno probabilmente tolto ossigeno allo scalo milanese ma che in assoluto non possono essere considerati un male in sé. Nel capoluogo lombardo l'aggravante è costituita, com'è stato ricordato, anche dall'incapacità di sfruttare l'occasione di un grande evento come l'Expo 2015, che dovrebbe costituire la straordinaria occasione di rilancio di queste dotazioni e che invece vede questo Governo latitare dalle proprie responsabilità. Ancora una volta è inevitabilmente la mancanza di una visione nell'azione di Governo che avvilisce la condizione degli scali nella mancanza di una politica coordinata. Ognuno di essi vive nel proprio localismo, relegato in asfittiche dinamiche di mercato dove la competizione non è di sistema e, quindi, rivolta verso l'esterno, ma è conflittuale perché orientata all'interno del Paese e, quindi, implosiva nella prospettiva. Occorre, allora, favorire una maggiore complementarietà degli scali sviluppandone e favorendone specializzazioni e vocazioni proprie di ogni territorio. è la differenza sostanziale di una politica che governa avendo un progetto in grado di orientare e regolare le dinamiche di mercato da una che si propone semplice dì favorirlo lasciandone liberi gli istinti e propugnandone una naturale selezione darwiniana che fa strame dei che fa strame dei soggetti più deboli, ma che non consente neppure ai più grandi di affermarsi. I risultati, come questa crisi dimostra, sono sotto gli occhi di tutti, crisi che contrariamente ai proclami di ottimismo non finisce, ma come vediamo anche oggi si avviluppa su sé stessa, confermando ancora di più la necessità di un'azione di Governo che sia davvero orientata all'interesse generale e alla tutela dei diritti dei singoli cittadini. Interesse generale che non è componibile con nessuna sommatoria degli interessi particolari, ma dalla sola sintesi che un'azione di governo deve proporsi, cosa che questo Governo, come è sempre più evidente, non è in grado di fare. Castelli, con la nostra mozione in fondo vogliamo spronarvi a fare proprio il vostro dovere: governare nell'interesse del Paese e a tutela dei diritti dei più deboli, i lavoratori *in primis*.

un tema che ovviamente implica una riflessione sull'intero sistema del trasporto aereo prima di entrare nello specifico di Malpensa. La storia di questo aeroporto nasce negli anni Ottanta, e nasce prevalentemente in una visione europea legata ad aeroporti visti come sistema *hub*, di un sistema di trasporto aereo che mirava a concentrare le destinazioni in un unico punto, in maniera tale da accumulare una quantità di traffico che poi venisse da quel punto rilanciata in una rete internazionale: un serbatoio di accumulo dei voli nazionali o internazionali di corto raggio, che diventasse un punto di rilancio nel medio-lungo raggio.

all'inizio degli anni Duemila, dopo il lavoro del gruppo di alto livello e dopo il lavoro del semestre italiano con Van Miert, è sfociata nella *quick short list* e quindi nel sistema dei corridoi europei,

5, Lisbona-Kiev, dal corridoio Genova-Rotterdam e dal corridoio Berlino-Palermo, l'aeroporto di Malpensa appare come un punto fondamentale, servito da questi corridoi, di cui a sua volta può usufruire là dove usufruire là dove è punto di destinazione. Quindi Malpensa, all'interno di questo quadro, vede confermato il suo ruolo. Ma che cosa ancora è cambiato da quel periodo?

è cambiata la logica del trasporto aereo, con il sistema cosiddetto *point to point*,che si è materializzato prevalentemente, anche se non esclusivamente, nel sistema *low cost*.

perché la quantità di trasporto aereo che è stata sottratta ai sistemi *hub* per effetto dei sistemi punto-punto viene recuperata, per effetto del sistema *low cost,* nella quantità di traffico complessivo del trasporto aereo, che non solo è aumentata in questi anni, ma che è prevista in fortissimo aumento nei 10-20 anni prossimi, fino ad arrivare addirittura, in alcune previsioni che possiamo anche considerare ottimistiche, nel decennio 2020-2030 a 100 milioni di passeggeri sia per l'aeroporto di Malpensa, sia per quello di Fiumicino. Fiumicino. È giusto quindi che vediamo l'aeroporto di Malpensa come il motore e il centro di un servizio indispensabile, di tutto

che ci occupiamo di verificare e controllare se le decisioni

nei tre anni trascorsi dall'ultima discussione, alcuni passi avanti siano stati fatti, sia sul sistema del trasporto aereo, sia su Malpensa. fatto anche negli interventi precedenti - parliamo di apertura di nuove vie di comunicazione nei confronti di Malpensa, sia delle ferrovie del Nord sia dei tratti stradali e autostradali, e comunque è previsto un ulteriore potenziamento di questo sistema di collegamenti in previsione dell'Expo 2015. il tratto sarà compiuto quando vi sarà un collegamento, il più possibile efficace ed efficiente con il sistema dell'alta velocità e quando il sistema dell'alta velocità sarà completo completo all'interno del corridoio 5 e del terzo valico e quindi del corridoio Genova-Rotterdam. Credo che ciò sia centrale nell'ottica della discussione che stiamo facendo su Malpensa, come servizio essenziale di tutto il sistema settentrionale del nostro Paese. Sotto questo profilo, le discussioni di questi mesi e di questi anni sul ruolo di Alitalia, sul sistema del trasporto aereo per quanto riguarda i vettori, sembrano ormai archeologia politica e industriale. Abbiamo accantonato tutta una serie di paure che riguardavano l'aeroporto di Malpensa e sono state prodotte una serie di azioni, chieste anche da questo Parlamento, soprattutto in ordine agli accordi bilaterali fra i vari Paesi. È per questo quindi che, ritenendo non nelle premesse, ma nella sostanza, molto simili le mozioni fra di loro,

con cui abbiamo cercato di raggiungere un'intesa per un testo unico che ha visto la condivisione massima sugli impegni al Governo, ma partendo da premesse